Onorevoli colleghi, in questi giorni ricorre il cinquantesimo anniversario dei fatti d'Ungheria. L'insurrezione di Budapest, con manifestazioni, scontri e coinvolgimento di studenti, operai e cittadini, ebbe conseguenze drammatiche per la vita di quel Paese. L'intervento del Patto di Varsavia causò 2.800 caduti. al di là di ogni visione ideologica, culturale, delle nostre storie e delle nostre divisioni, in senso buono, anche politiche, mi appare indubbio - e voglio sottolinearlo che un popolo insorse a difesa e a recupero della propria libertà e pagò questo con un durissimo prezzo di sangue.

credo che non sia azzardato rilevare tutti, con rammarico, che la dura divisione dell'Europa in due blocchi, così come si configurava nel 1956, impedì alla generosità, al coraggio, alla voglia di libertà di quel popolo di ottenere il successo che avrebbe meritato. Ricordo che il Senato - quindi noi - ha patrocinato l'iniziativa dell'università «La Sapienza» di Roma per una giornata di studio e memoria, il 7 novembre, con la partecipazione, tra gli altri, del Presidente della Repubblica di Ungheria. In ricordo dei caduti, di questa pagina forte in difesa della libertà dei popoli, vi invito ad osservare un momento di raccoglimento.

l'urgenza di calendarizzare il disegno di legge recante: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione della donna di origine extracomunitaria presente in Italia». Le vicende di questi ultimi giorni (e a tale proposito esprimo solidarietà alla collega della Camera, onorevole Santanchè, per quanto è avvenuto nella trasmissione televisiva che tutti abbiamo visto),

che hanno visto l'uccisione di una ragazza che voleva semplicemente avere un fidanzato italiano e uno uno stile di vita italiano, oppure gli episodi più grotteschi dell'*apartheid* al contrario di alcune facoltose donne musulmane che hanno potuto farsi riservare una spiaggia, in quel di Rimini,

molto brevemente per ricordare che nei giorni scorsi, sulla stampa della Campania e sulla stampa nazionale, abbiamo letto notizie circa minacce gravi e serie ad un magistrato della Direzione distrettuale antimafia. Vi è un'indagine in corso: tali minacce provengono dal *clan* dei Casalesi, e cioè da quella parte della camorra della Campania che fa centro su Caserta. Si tratta di un'organizzazione camorristica strutturata in modo verticistico, sul modello di Cosa nostra, capace di dominare il territorio. Già nei giorni scorsi vi erano state minacce ad uno scrittore per aver scritto un libro, che ha un qualche successo, che riguarda la camorra, e in particolare quella del casertano. Presidente di adoperarsi affinché il Governo venga a riferire sulla situazione nella provincia di Caserta, a Casal di Principe, sul significato e sulla gravità di queste intimidazioni e sulle misure che intende assumere per fronteggiare e combattere la minaccia camorristica.

in merito ai fatti che sono avvenuti in questi giorni e che hanno riguardato una nostra collega della Camera, intendo associarmi alle osservazioni che sono state fatte da due Ministre - la Pollastrini e la Turco che hanno proposto di costituire una commissione mista di donne di origine italiana e di donne di altre religioni (in modo particolare musulmane) affinché, anche all'interno del nostro Paese, si apra un confronto serio, franco e onesto, così da evitare forme di discriminazione. Voglio ricordare che la nostra legislazione prevede per i cittadini e le cittadine italiane, per una questione d'identità e di sicurezza, l'obbligo di mostrare il viso; possono però portare coperti la testa e i capelli. Credo che questo sia un elemento di incontro e non di divisione nei confronti di persone provenienti da etnie, religioni e culture diverse.

che in quest'Aula ci si soffermi per un attimo su quanto sta avvenendo in Ungheria in questi giorni e in queste ore. In un clima rarefatto, surreale si è svolta ieri a Budapest la cerimonia per celebrare il cinquantesimo anniversario di quella rivolta anticomunista. nelle stesse ore in cui lo si celebrava a livello istituzionale, senza la presenza del popolo (perché è stato impedito alla gente di accedere alla piazza del Parlamento dove si svolgeva la celebrazione),

lo stesso problema per dare poi una risposta adeguata. Al senatore Massimo Brutti comunico che ci faremo promotori di un intervento presso il Governo perché si venga a rispondere sul fenomeno della camorra, in particolare per Casal di Principe. Debbo dire - mi associo alle riflessioni del senatore Novi - che il momento è difficile anche in questi giorni in Ungheria ed è difficile per l'Europa. Abbiamo una ragione in più per intervenire: impegneremo il Governo italiano a chieder conto proprio della situazione di forte tensione che c'è in Ungheria.

all'unanimità modifiche ed integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori per il periodo dal 7 al 9 novembre, ovvero la settimana immediatamente successiva alla sospensione dei nostri lavori. Oggi pomeriggio saranno esaminati i disegni di legge recanti rendiconto e assestamento del bilancio dello Stato. Domani mattina inizierà la discussione del decreto-legge sul disagio abitativo, con i lavori della Commissione conclusi. Al termine della seduta antimeridiana di domani si passerà alle votazioni a scrutinio segreto sulle dimissioni reiterate dei senatori Bubbico e Pinza. Nel corso della seduta antimeridiana di giovedì 26 ottobre saranno discusse, oltre alla mozione sui flussi migratori, primo firmatario il senatore Mantovano, già prevista, le mozioni sulla Conferenza di Nairobi. Per tali documenti si è proceduto all'organizzazione delle rispettive discussioni: 15 minuti per ciascun Gruppo per la mozione sui flussi migratori, 10 minuti per Gruppo per la mozione sulla Conferenza di Nairobi. Il calendario della settimana prevede inoltre il disegno di legge, con procedura abbreviata, recante istituzione di una Commissione governativa di indagine sull'anziano. È stato poi rinviato alla seduta antimeridiana di giovedì 9 novembre, su richiesta del Governo, l'incardinamento della legge comunitaria 2006. Resta confermato che l'Assemblea non terrà seduta la prossima settimana, laddove le Commissioni potranno invece convocarsi in relazione ai rispettivi programmi di lavoro. Nella seduta antimeridiana di martedì 7 novembre avrà inizio l'esame del disegno di legge di riforma degli esami di istruzione secondaria superiore - ove definito, spero di sì, dalla Commissione - il quale potrà proseguire a conclusione dei decreti-legge in scadenza. A partire dal pomeriggio del 7 novembre saranno discussi i decreti-legge in materia di funzionalità della pubblica sicurezza e di emergenza rifiuti in Campania, per i quali i tempi sono stati ripartiti tra i Gruppi. Il calendario potrà essere integrato con l'esame delle proposte della Giunta per il Regolamento in tema di integrazione del Consiglio di Presidenza del Senato. Per quanto concerne il *question time* sui diritti umani in Cina,

Ritengo che dobbiamo denunziare il fatto che questa discussione generale sta dando la possibilità al Governo di recitare la seconda puntata di una storia stranamente farsesca. È una farsa farsesca. È una farsa a puntate: la prima puntata ha avuto luogo con la discussione del Documento di programmazione economico-finanziaria, la seconda puntata della farsa della manovra e della preparazione del bilancio 2007 il Governo la sta recitando oggi in quest'Aula. Perché è una farsa? Perché il Governo continua ad avere atteggiamenti stravaganti, condisce il suo operato con un certo realismo, cerca di mostrare storie ed eventi quotidiani, ma lo fa sempre in modo grottesco e irrazionale. In verità, dice cose che hanno configurazioni di verosimiglianza, ma poi aggiunge troppa, davvero troppa fantasia al suo operato. Parlo di troppa fantasia perché il Ministro dell'economia si è presentato al Parlamento e ha detto che l'Italia è in una situazione disastrosa, che la situazione è paragonabile soltanto a quella del 1992; poi corregge, con l'assestamento presentato in quest'Aula, i suoi stessi dati, corregge le entrate e nel farlo dice il vero, ma poi confonde le idee mischiando la nozione e la notizia rispetto all'aumento delle entrate con troppa fantasia.

le funzioni del rendiconto - così come assegnate dalla tradizione, ma ancor più come disposto della legge di contabilità - implicano la necessità di una valutazione amministrativa (cioè, i risultati si valutano sotto il profilo della gestione),

La valutazione di tipo politico sta nel fatto che il Parlamento deve valutare se il Governo ha perseguito correttamente gli obiettivi che erano stati fissati con la legge di bilancio di cui al rendiconto. Quindi, tutte le osservazioni che la maggioranza fa su una legge, il rendiconto, che ha una sua importanza di tipo formale, lasciano il tempo che trovano; è sull'assestamento che invece dovremmo correttamente parlare. Sull'assestamento dovremmo individuare quelle che sono le azioni politiche del Governo e non cercare di far refluire il dibattito sul rendiconto, ancorché è sull'assestamento che il Governo sta recitando la sua seconda puntata farsesca. Perché si tratta di una farsa? Perché

registra un aumento di entrate di 7 miliardi di euro. È una situazione che quindi lascia vedere come quello che si è fatto con le leggi finanziarie precedenti ha di fatto rilanciato l'Italia, ha dato la possibilità di cogliere un momento di ripresa; e la circostanza che sia stato colto il momento della ripresa

di dettare la necessità al Governo e al Paese di sopportare manovre di lacrime e sangue, aumento delle tasse e, conseguentemente, capitali che vanno via, *rating* che si abbassa. Basterebbe soltanto quell'effetto di Visco sul fisco e, invece, non è così, perché l'effetto sul fisco è stato determinato da un'azione corretta del precedente Governo nel perseguimento degli obiettivi che erano stati indicati nelle precedenti leggi di bilancio. Ma c'è una cosa in più che bisogna cercare di individuare, di capire e farsi spiegare dal Governo: perché nell'assestamento di bilancio aumenta l'autorizzazione all'emissione di BOT da 60.000 milioni di euro a 66.500, cioè 6.500 in più, più del 10 per cento di aumento nell'autorizzazione all'emissione di titoli. Questo non era mai avvenuto, salvo che nel 1995 e nel 1998, con Governi che non erano di centro-destra, cioè nel 1995 con il Governo Dini (e comunque aveva un significato, perché c'era stata una disarmonia nella conduzione della cosa pubblica) e nel 1998 per effetto dell'entrata nell'Unione Europea. Ma perché oggi, quando per tanti anni l'autorizzazione all'emissione di BOT è stata fatta in modo prudenziale? Non si capisce cosa stia avvenendo; se aumentano le entrate di 7 miliardi di euro, perché dare l'autorizzazione al Governo di emettere più Forse - ed è bene che questo resti agli atti parlamentari, perché così ha dichiarato il Governo in Commissione - per poter dare la possibilità al Governo di

Dice il Governo che tali emissioni sono compatibili con il limite delle emissioni nette sancite nella legge finanziaria del 2006. Allora, perché questo aumento nell'assestamento?

perché non riusciamo a capire l'esatta portata di quanto il Governo prima dichiara in Commissione e poi non fa con l'assestamento. Dice il Governo che si riserva di farlo per atto amministrativo. E perché procedere per atto amministrativo per un'entità così importante? Perché il Governo non opera oggi le giuste, naturali e opportune correzioni, dandoci la possibilità di vedere ciò che effettivamente succede, vale a dire di cogliere la realtà sostanziale del Presidente)*, che non ha bisogno di una manovra da 40 miliardi di euro, ma che avrebbe bisogno di una manovra molto molto più contenuta? In tal modo, infatti, si sarebbe realizzata nel Paese una conduzione più seria e più opportuna.

i dati sono evidenti e, se questa fosse una favola, potremmo cominciare da: «C'era una volta». Per il «c'era una volta» potremmo ricordare la commissione Faini

le agenzie potrebbero abbassare il *rating*. Per fortuna, però, il tecnico Padoa-Schioppa ci aveva raccontato che, grazie al suo intervento, le agenzie di *rating* si erano convinte e avevano mantenuto il livello di fiducia nel nostro Paese. La favola purtroppo non è finita bene: le agenzie di *rating* non solo non hanno creduto al ministro Padoa-Schioppa, non hanno creduto al provvedimento Bersani-Visco, il primo provvedimento vampiresco che avete messo in atto (il secondo lo state facendo adesso) e hanno abbassato il grado di fiducia nel Paese. Certo, se lo avesse fatto il Governo Berlusconi sareste insorti o quant'altro. di vista politico questo assestamento di bilancio e quindi, come ha già detto il collega Ferrara, la farsa dei conti pubblici, basta citare

l'IRPEF ha registrato una crescita del 6,4 per cento. Ci dite poco! Se adesso state cercando di rivedere in qualche modo la manovra finanziaria, lo fate perché c'è una dotazione di cassa che proviene dalla scorsa finanziaria

ma avete anche contribuito, con la commissione Faini, a creare un generale malcontento-scontento punito dalle agenzie di *rating*. con l'assestamento, troviamo solamente 6 miliardi di maggiori entrate, visto che nei primi otto mesi le entrate superano i 25 miliardi per ammissione stessa

del Governo, quest'oggi relazioniamo in merito a un rendiconto e a un documento di assestamento le cui variazioni, che si aggiungono ad altre già effettuate per atto amministrativo, incrementano il saldo netto da finanziare per il 2006 da 36.664 milioni di euro a 38.464 milioni. Il saldo primario resta positivo, ma scende da 34.736 milioni di euro a 33.229 milioni. Il ricorso al mercato dovrebbe aumentare da 232.666 milioni di euro a 235.595 milioni. Questi sono i numeri fondamentali dei due provvedimenti che ci accingiamo a votare. Tale peggioramento è da porre in relazione all'andamento delle spese finali, soprattutto delle spese correnti primarie, che registrano un incremento solo parzialmente bilanciato dal miglioramento delle previsioni relative alle entrate finali. Il documento di assestamento, peraltro, registra la crescita delle entrate finali, un aumento, già nel testo presentato il 30 giugno, di circa 2.200 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali di bilancio. Con un emendamento presentato dal Governo a settembre le entrate sono state ulteriormente corrette verso l'alto per circa 10 miliardi. In particolare, l'IRE cresce di 3,6 miliardi di euro e l'IRES di 2,5 miliardi di euro. Le imposte sostitutive, già segnalate in crescita di 900 milioni a giugno, registrano una previsione complessiva di più 3,4 miliardi. L'IVA sugli scambi interni ed intracomunitari cresce di ulteriori 2,1 miliardi, mentre l'IVA sulle importazioni di ulteriori 1,15 miliardi. Questi sono i numeri che danno la fotografia esatta di un rendiconto, già presentato in Commissione bilancio, dove gli esponenti della Casa delle Libertà hanno sottolineato come alla grande drammatizzazione mediatica sullo stato dei conti pubblici, attuata dalla sinistra subito dopo le elezioni, sia poi seguito un implicito riconoscimento che il miglioramento strutturale delle entrate, dovute a buone politiche, sia dovuto alle attività del Governo Berlusconi. La Casa delle Libertà ha infine chiesto un'operazione verità sulle condizioni di finanza pubblica e il vostro Governo ha dovuto ammettere, come altri colleghi hanno segnalato

e un rapporto sotto il segno della trasparenza e della responsabilità con i cittadini. Altro che evasori fiscali, sono cittadini che lavorano ogni giorno, che producono quanto di buono c'è in questo Paese e che vanno trattati come meritano *(Applausi questo Paese ogni mattina, alzandosi presto e lavorando, malgrado noi, malgrado l'attività che spesso questo Parlamento non riesce a svolgere nel migliore dei modi quando deve rappresentare le loro istanze. Non esiste quindi una tassa di successione dei presunti guasti del Governo Berlusconi di vischiana memoria, questo Visco che è una grande sciagura per il nostro Paese. Resti agli atti del Parlamento, invece, che il Governo Berlusconi ha lasciato buone politiche di sviluppo economico ed occupazionale, come ha ricordato bene il collega Polledri, e conti pubblici in buono stato, mentre a questo Governo sono bastati pochi atti, a partire dal cosiddetto decreto Visco-Bersani, per raccogliere giudizi pesantemente negativi dai mercati internazionali, fino al clamoroso declassamento dell'Italia da parte delle agenzie di *rating*. Voi continuerete su questa strada, ne siamo certi. Noi speriamo di riuscire a fermarvi, ma ci consoliamo pensando che fra trent'anni - come avviene per i fatti di Budapest che in questi

Signor Presidente, colleghi senatori, colleghe senatrici, il rendiconto - come spero sia emerso chiaramente dalla relazione - descrive una situazione economica e finanziaria per l'anno 2005 critica e deficitaria. del dibattito, peraltro sintetico, sono state ribadite interpretazioni politiche anche divergenti, rispetto a quelle presentate dalla relazione. Non ci sono state però proposte emendative per ciò che concerne il rendiconto, quindi non mi resta che confermare un giudizio critico sui conti dello Stato per l'anno finanziario 2005

la mia replica sarà brevissima, perché gli argomenti emersi dalla discussione generale in realtà non cambiano lo scenario che abbiamo davanti.

e della spesa primaria, in particolare per l'anno 2006. Rimane pertanto confermata la necessità di operare in modo rigoroso, facendo tesoro anche delle maggiori entrate tributarie che sono state accertate e che

Signor Presidente, onorevoli senatori, la discussione che si è svolta in Aula

con i quali il nostro Paese si deve misurare, che riguardano in maniera specifica la situazione dei conti pubblici. Voglio riprendere, in maniera molto rapida, alcuni dei temi di particolare delicatezza con i quali ci troviamo a misurarci e di cui abbiamo già dato conto in sede di aggiornamento del DPEF e nel corso della discussione che si svolge in occasione della predisposizione dello strumento finanziario per il 2007. una situazione che ha visto crescere, contrariamente alle indicazioni date, la spesa corrente, che ha visto una riduzione degli investimenti, tanto che siamo stati costretti, nella siamo stati costretti, nella fase precedente all'assestamento, ad una manovra correttiva per finanziare cantieri ed infrastrutture. In maniera identica, si è intervenuti in fase di assestamento su alcune altre voci. Per il resto occorre sottolineare le novità più rilevanti della discussione che riguardano un aumento delle entrate che, però, sono compensate negativamente dalla sentenza della Corte europea in materia di In conclusione del mio intervento, voglio confermare per intero la volontà del Governo di perseguire come obiettivo principale quello del risanamento dei conti pubblici e, in maniera congiunta, operare per un rilancio della competitività del nostro Paese. Non è casuale, a questo proposito, la grande attenzione che è stata posta nella proposta di legge finanziaria al tema della competitività delle imprese, e quindi al loro sostegno e alle risorse da destinare allo sviluppo. Una sola precisazione rispetto al tema sollevato senatore Ferrara: relativamente all'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, vorrei ricordare che quella previsione era contenuta come obiettivo nella trimestrale di cassa del 31 dicembre 2005. Abbiamo confermato tale previsione, ma l'orientamento del Governo, ovviamente, è quello di non far ricorso alla massima espansione dei titoli.

Comunico che, poiché la votazione finale del rendiconto così come quella dell'assestamento avverrà mediante scrutinio elettronico, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, una volta concluso l'esame degli articoli del rendiconto, si passerà direttamente alla discussione degli articoli dell'assestamento. Seguiranno poi le dichiarazioni di voto congiunte e avranno, quindi, luogo le due votazioni con il sistema elettronico. Procediamo pertanto all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1059. Passiamo

ai fondi per la ricerca scientifica, ai fondi per le aree sottoutilizzate e ai fondi

dell'appostazione, in sede di assestamento, di due minori entrate che sono state accettate puntualmente dal Governo e riportate nella Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico‑finanziaria.

per ciò che riguarda gli anni passati e per 3 miliardi e 700 milioni di euro per quanto riguarda il presente. Si è sostenuto, in sede di Commissione bilancio,

ammontare di una finanziaria, cioè 13 miliardi e 400 milioni di euro per il passato e 3 miliardi e 700 milioni di euro a regime, è una tesi molto ardita, azzardata e che comunque sottrae al Parlamento la decisione su una materia finanziaria di così grande rilevanza. Molto banalmente comprendo che il Governo non intende modificare il disegno di legge di assestamento solo perché non vuole portarlo in terza lettura ma francamente questa mi sembra una tesi ancor più banale. Non parliamo, signor Presidente e colleghi, di piccole somme, ma di 13 miliardi e 400 milioni di euro e di 3 miliardi e 700 milioni di euro.

vulnerata da un atteggiamento negativo del Governo e della maggioranza.

una prima considerazione generale sugli emendamenti proposti. Come bene ha rilevato il senatore Azzollini, alcuni degli emendamenti presentati sono il segno di scelte di politica economica.

Quanto alla questione relativa al mancato recepimento degli effetti della sentenza europea in materia di IVA ed ai relativi emendamenti presentati, è pacifico che nella nota di aggiornamento del DPEF il Governo ha quantificato l'impatto negativo sul gettito per il 2006 e quello, in ragione della competenza economica, per la corresponsione degli arretrati. Anche in forza del recente decreto‑legge già convertito avente ad oggetto proprio tale questione, il Governo ha precisato che non si prevedono corrispondenti variazioni ai fini del saldo netto da finanziare di competenza e di cassa relativo all'anno 2006, questo in considerazione dei diversi criteri di contabilizzazione di tali poste che, ai fini dell'assestamento in esame, vedono previsioni costruite in termini di contabilità finanziaria mentre, correttamente, nella nota di aggiornamento del DPEF sono state formulate in termini di competenza economica. Si esprime, pertanto, parere contrario su tutti

Preso atto del ritiro degli emendamenti presentati dal senatore Legnini, confermo il parere contrario su tutti i rimanenti emendamenti per le ragioni appena descritte. Quanto all'ordine del giorno G100 presentato dalla sottoscritta, non mi dilungo

della Commissione bilancio il parere per la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF di pertinenza statale per il 2006 e, vista l'esiguità delle risorse rimaste a disposizione, a fronte di 1.601 domande-progetto presentate per finalità

a disporre, fin dalla legge finanziaria per l'anno 2007, l'integrale ripristino della quota dell'otto per mille dell'IRPEF di pertinenza statale ovvero, in ogni caso, ad assicurare la piena destinazione di queste risorse alle finalità sociali, culturali e umanitarie proprie di tale istituto», attuazione e rispettare le indicazioni che sono state espresse dai cittadini contribuenti al momento dell'esercizio dell'opzione. Quanto all'ordine del giorno G1.100, presentato dal senatore Legnini, la relatrice esprime parere favorevole.

gli effetti della famosa sentenza sull'IVA. La somma dei due emendamenti - faccio presente alla maggioranza e alla minoranza - ha come entità complessiva la metà dell'importo della manovra finanziaria per l'anno 2007;

ma necessario per il raggiungimento degli obiettivi di rigore, che ritengo debbano essere supportati adeguatamente da qualsiasi Governo, non soltanto di quello

debito pubblico per 66,5 miliardi di euro è soltanto una pura ipotesi di lavoro. Non si fanno i bilanci con le ipotesi di lavoro; i bilanci si fanno con i dati reali, con il rigore dei conti.

e, contemporaneamente, non inserire tali cifre nell'assestamento di bilancio. Ma la cosa ancor più grave è che di fatto il Governo le ha previste perchè nella prima seduta farsesca, quella relativa al Documento di programmazione economico-finanziaria, i dati sono stati registrati. Infatti, oggi l'indebitamento non sarebbe quello dichiarato dal Governo nella Nota se non ci fossero gli effetti della sentenza IVA, il debito non sarebbe quello dichiarato nella Nota se non ci fossero gli effetti della sentenza IVA, e allora questi effetti ci sono o no? Non possono aleggiare nei conti dello Stato. Ci vuole chiarezza e rigore. Con gli

lavori, faccia amministrazione e politica con la realtà di bilancio. Questo bilancio non è reale e neanche assestato. Questo assestamento è sostanzialmente - mi scusi la forzatura della parola - falso. Noi siamo contro la falsità e chiediamo di approvare questo emendamento.

all'emendamento 1.Tab.1.1) sottrarrebbe al Parlamento nazionale - cari colleghi, questo è stato sostenuto - la decisione su ben 13 miliardi e 400 milioni di euro. sottrarrebbe al Parlamento nazionale, per affidarla ad un atto amministrativo del Governo, la decisione circa il governo, dal punto di vista finanziario, degli effetti della nota sentenza della Corte di Bruxelles a proposito dell'IVA sulle automobili delle imprese. Tanto, infatti, il Governo, sulla base di relazioni tecniche approntate per altri provvedimenti, ha valutato che sia l'effetto determinato da quella sentenza sui conti pubblici italiani. Naturalmente - lo dico per coloro che stanno ascoltando questa discussione - i 13 miliardi e 400 milioni di euro si riferiscono al complesso delle conseguenze circa il pregresso

Signor Presidente, io sostengo che non è affatto fondata la tesi, a sua volta sostenuta dal senatore Azzollini, secondo cui cui il Governo darebbe parere contrario e la maggioranza si esprimerebbe in maniera contraria a questi emendamenti sulla base della mera esigenza di non fare una terza lettura alla Camera (cosa che risulterebbe necessaria se quest'Aula approvasse uno o più d'uno di questi emendamenti). Il fatto è,

La ragione, signor Presidente, ha qualche complessità tecnica, ma è quasi impossibile parlare di cose così complicate in un contesto di questo tipo... ammesso che ci sia qualcuno che voglia seguire questa discussione che sembra riguardare, e riguarda effettivamente, qualcosa come più di 25.000 miliardi di vecchie lire, la questione

ed è stata invece pagata dai soggetti indicati dalla sentenza, per 13 miliardi e 400 milioni di euro. e 400 milioni di euro. Voi sapete, signor Presidente, colleghi, che esistono due tipi di contabilità: una è la contabilità economica, quella in base alla quale, su valutazioni di competenza giuridica, si determina il dato del cosiddetto indebitamente netto delle pubbliche amministrazioni in rapporto al prodotto interno lordo (quello che vale per il Patto di stabilità esterno e per Bruxelles); è poi un dato relativo invece a qualcosa che ha più a che fare con la cassa che con la competenza, ossia il dato del fabbisogno e, di conseguenza, del saldo netto da finanziare. Ora, in termini di SEC 95, cioè sulla base delle regole di contabilità europea, è chiarissimo che lo Stato italiano debba contabilizzare, in termini di contabilità economica, così peggiorando il dato dell'indebitamente netto

cioè nell'anno in cui si determina l'obbligazione a pagare, o, come in questo caso, l'obbligazione a restituire ciò che è stato, secondo la sentenza, Così il Governo ha fatto quando, nella Nota di aggiornamento al DPEF, ha registrato il peggioramento per un punto e qualcosa di PIL del dato dell'indebitamento netto.

ai soggetti interessati dalla sentenza di recuperare le somme illegittimamente pagate, in quel momento sarà registrato un dato negativo sul piano del fabbisogno e a quel punto la contabilità finanziaria dovrà registrarlo, cosa che puntualmente la legge finanziaria per il 2007 e per gli anni successivi fa, determinando le conseguenti variazioni nella legge di bilancio. È del tutto evidente - e termino, signor Presidente - che se nel 2006 materialmente non viene erogato nulla, in termini di fabbisogno il dato di peggioramento dei conti è certamente pari mentre il dato di peggioramento dell'indebitamento è di 13 miliardi e 400 milioni. Come deve essere registrato nei dati di contabilità nazionale un tale peggioramento dell'indebitamento? In termini di

perché si tratta di un evento esterno all'attività di legislazione, cioè di una sentenza della Corte di Bruxelles che scarica degli oneri sulla finanza pubblica italiana. È il caso classico nel quale

l'intervento del senatore Morando in ordine alla contrarietà, espressa per voce sua dalla maggioranza, all'approvazione dell'emendamento sui 13,4 miliardi di euro

Volendo continuare nella logica del ragionamento, il Governo su questo emendamento ha dato parere contrario perché ritiene che, non essendo ancora certi gli esiti, non si debba preoccupare dell'assestamento della relativa cifra, con effetti sul bilancio del 2006. Ma se così fosse e se quindi avesse validità il ragionamento del senatore Morando, significherebbe che, per lo spazio temporale intercorrente tra il 14 settembre e la fine dell'anno, non dovrebbero esserci effetti della cosiddetta sentenza IVA sulla richiesta di detrazione dell' IVA pagata nell'acquisto degli automezzi. Ma così non è, tant'è vero che non solo nel Documento di programmazione economico-finanziaria era stata scontata la cifra di 3,7 miliardi in funzione dell'indebitamento, ma che in tutte le dichiarazioni si dice che sui 3,7 miliardi di euro sarà fatta compensazione durante l'anno.

il Governo presenta il suo emendamento alla Camera dei deputati, si chiarisce che la proposta di assestamento per 2,132 miliardi - che era la previsione iniziale - andava corretta di 4,8

lire. Ripeto, il Governo non ci dice se la sua contrarietà all'approvazione dell'emendamento derivi dal fatto che non ci sarà l'esborso di 3,7 miliardi di euro o se invece, nonostante l'esborso, non ci voglia dire se l'assestamento deve essere fatto

*(LNP)*. Signor Presidente, proprio contestualmente all'istituzione di una Commissione d'inchiesta sul lavoro nero nel mondo agricolo, soprattutto nel Meridione, l'emendamento 1.Tab.2.4 consente di fornire finanziamenti alle forze dell'ordine, al fine di consentire loro di operare controlli e di reprimere questa piaga. Quindi, trovo giusto che l'emendamento 1.Tab.2.4 sia votato in modo positivo da quest'Aula; mi spiace che sia stato ritirato dal presentatore, lo facciamo nostro e chiediamo all'Aula di non togliere finanziamenti che servono per l'acquisto anche di automezzi, magari sostituendo le vecchie FIAT «Uno», che credo siano ormai neppure euro, sono

Signor Presidente, onorevoli senatori, intervengo su entrambi i provvedimenti, rendiconto del 2005 ed assestamento del 2006, la cui discussione è appunto congiunta. Come hanno avuto modo di rilevare diversi colleghi durante la discussione, i due documenti propongono un metodo di controllo tardivo e superato, che comporterebbe quindi una riscrittura della legge di contabilità pubblica e l'introduzione di sistemi più efficaci e puntuali. Dall'analisi degli stessi documenti e dal collegamento degli elementi di questi con gli altri documenti contabili appena presentati o approvati in Parlamento, si possono però rilevare dei dati di tendenza che evidenziano il quadro di come siano stati amministrati i conti pubblici negli anni in cui ha governato il centro-destra. Si tratta di anni che segnano, soprattutto nel periodo di fine legislatura, un aumento dell'indebitamento Il risultato differenziale tra le entrate e le spese finali decurtate delle operazioni finanziarie, che aveva avuto un *trend* decrescente fino al 2001 portandosi al 3,1 per cento, è tornato a crescere con i Governi Berlusconi, portandosi fino al 4,1 per cento registrato alla fine del 2005. Ciò soprattutto a causa di un forte aumento della spesa che non trova un corrispettivo nelle entrate. Dal punto di vista della spesa pubblica, si deve quindi annotare non solo un aumento della stessa, ma soprattutto una sua diversa e peggiore allocazione. Aumenta - anziché diminuire, come sarebbe auspicabile - soprattutto la spesa corrente. Si ingrandisce la spesa per quanto riguarda il pubblico impiego: ciò non significa che siano aumentati gli stipendi pubblici, ma che si è allargata la platea di chi ne di chi ne usufruisce, ossia sono aumentate proprio le voci dove invece si potevano introdurre dei controlli di spesa più rigorosi. Tali controlli sono mancati in generale, se ci troviamo a registrare, nei documenti in esame, delle eccedenze in molte voci di spesa che, per forza di cose, in quanto già impegnate, lo Stato deve onorare. L'aumento della spesa corrente è tutto a scapito di quella in conto capitale, cioè degli investimenti duraturi che avrebbero potuto segnare un serio cambio di marcia della politica economica e a favore dello sviluppo del nostro Paese. Se si considera che per ogni euro speso in conto capitale se ne spendono dieci per la parte corrente, avremo la misura di uno Stato che, purtroppo, è destinato a mancare importanti obiettivi di crescita, se non si mette in moto in tempi brevi una netta inversione di tendenza. Dal punto di vista delle entrate rileviamo come sia ancora troppo consistente, rispetto al totale delle entrate, il gettito da imposta sui redditi, in particolare da lavoro e, nella specie, e, nella specie, da lavoro dipendente. Noi riteniamo auspicabile una diversa distribuzione delle entrate; in particolare, pensiamo a minori imposte dirette compensate da maggiori imposte indirette. Secondo noi si può recuperare molta parte dell'evasione e dell'elusione fiscale attraverso la tassazione dei consumi e del trasferimento di ricchezza, perché solo in questo modo si possono colpire gli evasori e gli elusori fiscali ancor prima di attuare opportuni e appropriati controlli sui redditi. La revisione del sistema di tassazione da noi indicato, inserita in un quadro di perequazione generale, può portare soprattutto ad un graduale ed auspicabile abbassamento della tassazione sui redditi da lavoro negli anni a venire. La decisione dei Governi Berlusconi di puntare quasi tutto su misure *una* *tantum*, derivanti prima dalla cessione di parte del patrimonio pubblico e poi da condoni e scudi fiscali, ha creato danni sia alla gestione fiscale che al rapporto con i contribuenti ed ha lasciato in eredità ai Governi successivi gli evidenti limiti della mancata introduzione di interventi strutturali sulle entrate e sulle fiscalità. Crediamo che il Governo Prodi, a partire dal cosiddetto decreto Visco-Bersani ed ora con la manovra per il 2007, si stia muovendo nel senso di recuperare un rapporto con i contribuenti, con tutti, anche con quelli che sinora non sono stati onesti,

come previsto dalla vigente legge di contabilità. I disegni di legge in esame fotografano però il momento della gestione precedente, quella del centro‑destra, e indicano come ci si debba muovere di conseguenza. Ebbene, a noi sembra che il Governo Prodi e la sua maggioranza stiano puntando a una migliore qualificazione della spesa pubblica, ad una diversa e più equa gestione delle entrate, a obiettivi di finanza pubblica che possono portare il Paese a posizioni di crescita duratura, al fine di registrare nel giro di pochi anni un netto miglioramento dei conti pubblici. Per queste ragioni, dichiaro il voto favorevole sui disegni di legge in esame a nome del Gruppo che rappresento, i Popolari-Udeur, e - come vice presidente del Gruppo Misto, delegato dal

della situazione congiunturale, come spesso si fa, perché, mentre noi siamo stati fermi, l'Europa già l'anno scorso ha ripreso a camminare.

I numeri indicano inoltre che il debito pubblico è salito al 106,4 per cento

iniziando con l'ultimo passato Governo Berlusconi, il disavanzo dell'amministrazione pubblica ha perforato il limite che avevamo già sottopassato del 3,2 per cento, previsto dagli accordi di Maastricht. Il disavanzo è cresciuto fino al 2005 del 2,6 per cento del PIL. Per quest'anno si prevede un disavanzo pubblico del 4,6 per Il debito complessivo dell'amministrazione pubblica ha raggiunto il massimo storico del 100,6 percento del Prodotto interno lordo. Anche questa cifra dice poco. Cerco di esemplificare: immaginiamoci una famiglia, il cui debito è talmente grande che quello che si guadagna deve essere investito per pagare le rate e gli interessi alle banche.

Ho fatto questo quadro per far emergere le cifre e la situazione dell'Italia per un semplice motivo che riguarda la finanziaria futura. In tutta la discussione su questa finanziaria presentata dal Governo, si sentono solo interessi di parte. E soprattutto da certe categorie economiche sembra quasi che quel che conti per fare una finanziaria sia la somma degli interessi particolari di certe categorie. Invece siamo di fronte ad un debito pubblico talmente forte che deve essere nell'interesse di noi tutti e, soprattutto delle aziende e dell'economia tutta insieme, far crescere e far riprendere nuovamente questo Paese. Solo da queste cifre capiamo come, su una finanziaria di circa 40 miliardi, sarà prevista la manovra finanziaria prossima: quasi la metà sarà dedicata allo sdebitamento di questo peso, che si è accumulato soprattutto negli ultimi anni. anni. In questi ultimi anni, infatti, sul lato delle entrate, i continui e reiterati condoni fiscali, la legittimazione morale dell'evasione fiscale ha portato ad una economia sommersa di circa 200 miliardi di euro, che mancano e che devono essere pagati dai contribuenti che, invece, pagano onestamente le loro tasse. questo l'obiettivo di combattere questa evasione fiscale è più che plaudibile; non solo, è necessario per poter ridurre anche a lungo termine questo peso che sta gravando sulle spalle di chi lavora, sia come autonomo che come lavoratore per la nostra economia. Sono salite anche le spese correnti, nonostante i ripetuti vincoli formali posti per contenerle nelle leggi finanziarie che si sono succedute dal 2001 al 2005. Il dramma di questa situazione è che tale aumento delle spese correnti non è servito né a rilanciare l'economia né tantomeno a migliorare il livello dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni ai cittadini.

che serve una manovra finanziaria che abbatta il grandissimo *deficit*, un indebitamento dello Stato che non è più sopportabile. Ripeto l'esempio di una famiglia che, pagando tutto quello che guadagna esclusivamente per gli interessi, non ha più spazio per coprire

Ora, grazie alle vostre garanzie, ci troviamo con un quarto di punto e con qualche centinaio di milioni di euro in più da pagare! Quindi, avete raccontato al Paese

l'IVA sui consumi e quindi c'è meno "nero". Avete raccontato bugie al Paese e giustamente il ministro Padoa-Schioppa oggi non ha il coraggio di presentarsi in Parlamento. Per questi motivi molto semplici, consegniamo al Paese il voto contrario del Gruppo Lega Nord sui

il Gruppo dell'Ulivo voterà a favore dell'approvazione dei disegni di legge che stiamo discutendo, al fine di ottenerne una rapida definizione, necessaria al prosieguo della sessione di bilancio. Trattasi di strumenti, quelli del rendiconto e dell'assestamento, di contenuto prevalentemente se non esclusivamente tecnico-contabile, per i quali quindi l'esercizio della discrezionalità riconducibile a scelte di politiche di bilancio è contenuto entro margini molto ristretti, peraltro nel nostro caso non utilizzati in quanto il Governo ha sottolineato la necessità, e condividiamo tale posizione, di evitare una doppia lettura alla Camera, la quale conseguirebbe un inopportuno rallentamento della sessione di bilancio. Il nostro voto favorevole è quindi espressione di tali esigenze, prevalentemente tecniche, come detto, e legate all'ordinato svolgimento degli obblighi incombenti sul Parlamento. L'unica annotazione emersa sia nella discussione che nella discussione in Commissione che merita di essere evidenziata è quella che riguarda l'inadeguatezza di tali strumenti contabili rispetto all'esigenza di ottenere a consuntivo un quadro della gestione della finanza pubblica utile a verificare *ex post* il pieno rispetto degli obiettivi fissati dalla legge finanziaria e, in generale, degli strumenti di programmazione economico‑finanziaria. I documenti che dobbiamo approvare non consentono infatti di restituire al Parlamento, e quindi al Paese, un chiaro ed esaustivo quadro contabile contenente la misurazione a consuntivo degli obiettivi essenziali utili a valutare l'efficacia della gestione finanziaria dell'esercizio. Non consentono di valutare con immediatezza, ad esempio, il rispetto dei vincoli e delle regole del patto di stabilità esterno e in generale degli obiettivi di contenimento e controllo della spesa pubblica e delle entrate nel loro complesso e dell'incidenza delle politiche di bilancio sull'andamento dell'economia del Paese. Tale inadeguatezza non è evidentemente frutto di difetti compilativi del rendiconto e dell'assestamento, ma solo della struttura e della funzione di tali strumenti contabili, così come definiti e normati dalla legge di contabilità. È auspicabile che sul punto si avvii, come già si è fatto per il DPEF, una discussione in profondità per pervenire a uno sforzo riformatore risolutivo. Purtuttavia, l'occasione è utile per ribadire un giudizio per noi fortemente negativo sulla gestione finanziaria dell'anno 2005. Tale esercizio costituisce infatti il punto di caduta più basso delle politiche di bilancio del centro-destra del quinquiennio passato, l'anno nero dopo che in quelli precedenti le *performance* della finanza pubblica erano state nella migliore delle ipotesi deludenti. Signori dell'odierna opposizione, che fino a d'oggi, fino a poco fa, avete urlato supposti successi del vostro Governo e contestato i dati che vengono oggi riferiti dal Governo, i dati di cui abbiamo dovuto nostro malgrado prendere atto e sui quali siamo oggi costretti a ricostruire un quadro finanziario affidabile e accettabile del Paese per i mercati e l'Europa sono chiari e univoci. Il 2005 è stato l'anno nel quale si sono verificati, ad onta di illusorie e false previsioni, fatti che hanno compromesso l'accumulazione di credibilità

per un ammontare di enorme entità: il 2,8 per cento del PIL. Avete dilapidato le risorse in termini di cassa facendole aumentare dagli oltre 49 milioni di euro, cento del PIL del 2004, agli oltre 59 milioni di euro del 2005, il 4,2 per cento del prodotto interno lordo. Avete consumato l'avanzo primario che era stato con fatica e sacrificio ricostituito,

Per effetto delle incaute previsioni e della poco assennata gestione, il debito pubblico è balzato - come è stato detto - dal 103,9 per cento del PIL nel 2004 per cento nel 2005. A tutto ciò si possono aggiungere i dati notoriamente negativi dell'andamento dell'economia reale, causa ed effetto, almeno in parte, delle politiche di bilancio del Governo passato e l'inidoneità, evidenziata in tempi non sospetti dall'allora opposizione, di talune regole di contenimento della spesa: valgano per tutti gli esempi della regola del tetto del 2 per cento e dei tagli non selettivi ed indiscriminati espressi in termini percentuali sulla spesa dei Ministeri, tagli rivelatisi - come è noto - iniqui ed inefficaci. comincia ad essere completo. È un quadro che ci preoccupa, che è stato alla base di scelte molto impegnative che il Governo attualmente in carica ha programmato nel DPEF ed attuato nel disegno di legge finanziaria proposta al Parlamento. risultati che dovrebbero far riflettere voi, signori dell'opposizione, che dovrebbero indurvi ad un'autocritica severa e che, comunque, dovrebbero consigliarvi una maggiore cautela nelle posizioni politiche che andate esponendo

Prima di urlare nei modi che avete adottato e che state adottando anche oggi, prima di scendere in piazza e di assumere posizioni irresponsabili, dovreste riflettere, farvi carico dell'eredità che avete trasmesso al Paese e a chi oggi ha la responsabilità di governarlo. Ecco perché, signor Presidente, dietro i numeri che sostanziano i documenti contabili di assestamento e di consuntivo è nascosto un testamento che esprime tutte le difficoltà in cui si dibatte il nostro Paese, un testamento scritto da altri che, loro sì, hanno tradito la fiducia e le aspettative del Paese. È con questo spirito di grande preoccupazione, ma anche con la responsabilità e la determinazione necessarie per uscire in positivo da tale situazione, risanando, provando a reintrodurre una quota accettabile di giustizia sociale e a determinare le condizioni per far crescere di nuovo la nostra economia, che ci accingiamo a votare,

Signor Presidente, onorevoli senatori, membri del Governo, preliminarmente, ai fini di inquadrare meglio la situazione dei conti pubblici, giova rammentare che la Nota di aggiornamento al DPEF 2007-2011 appalesato come il PIL dell'anno in corso, nonostante le previsioni, sia in crescita, come le entrate fiscali siano maggiori e, soprattutto, come esse siano maggiori in maniera strutturale, il che significa che dispiegheranno i loro effetti anche l'anno prossimo. A questo punto, non vale pertanto neanche la pena di commentare ulteriormente la poco commendevole operazione attuata mediante la cosiddetta *due diligence* per il tramite di un economista pennivendolo, tant'è che ora lo stesso economista viene candidato a capo di varie commissioni di verifica dei conti pubblici (meglio sarebbe dire di inquisizione o di manipolazione dei conti), quali quelle create *ad hoc* dal disegno di legge finanziaria 2007. 2007. Venendo allo specifico dei documenti al nostro esame, rilevo come il dibattito in Commissione bilancio in ordine al rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2005 non abbia in alcun modo messo in discussione le risultanze di tale documento, che appare quindi sostanzialmente corretto, al di là delle ovvie differenze

per l'esercizio finanziario 2005 non abbia in alcun modo messo in discussione le risultanze di tale documento, che appare quindi sostanzialmente corretto, al di là delle ovvie differenze di valutazione tra maggioranza e opposizione. In proposito, faccio solo una notazione di sistema per rilevare come da tale documento non sia ancora del tutto possibile effettuare né la prevista valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti dagli indicatori di efficacia e di efficienza e agli scopi delle principali leggi di spesa, né il completo raccordo tra

Gruppo. Per quanto attiene, invece, al disegno di legge di assestamento per il 2006, non può essere sottaciuto, a mio parere, come le nuove e significative entrate che sono state oggetto di apposito emendamento presentato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati facciano ulteriormente giustizia della verità dei conti pubblici e della bontà della gestione di bilancio operata dal Governo Berlusconi. Su tale argomento, un elemento invece certamente censurabile è costituito dal fatto che è rimasta inevasa la questione della necessità di un di un approfondimento circa la natura di tali maggiori entrate ed in particolare sulla componente strutturale, ovvero congiunturale, delle medesime. Occorre infatti rammentare che la Nota di aggiornamento al DPEF stimava 5 miliardi di euro di maggiori entrate come componente strutturale, per cui appare chiaro come il migliore andamento economico non appaia da solo idoneo a giustificare l'intera entità delle maggiori entrate. Si può altresì affermare, come d'altronde emerso durante l'esame in sede di Commissione finanze della Camera, che parte della componente strutturale delle maggiori entrate potrebbe intendersi come effetto virtuoso dei condoni operati, che inducono molti contribuenti a dichiarare redditi sommersi favorendo un fenomeno di emersione dell'imponibile. Senza entrare nel merito di un dibattito che sarà affrontato in sede di esame del disegno di legge finanziaria 2007, mi sembra chiaro come, a partire dall'ingresso nell'euro, il Paese abbia pagato con una costosa fase di bassa crescita l'impreparazione con la quale si è entrati nel regime della moneta unica. Il bilancio pubblico ha dovuto pertanto necessariamente subire gli effetti di questo stato di cose. Ora esso deve imparare a muoversi in regimi di mercato veramente liberi e competitivi, creando le condizioni, le garanzie e le possibilità, per chi lavora e merita, di cogliere le opportunità, senza attendersi l'aiuto dello Stato. Signor Presidente, onorevoli senatori, membri del Governo, valutate tutte queste circostanze, non possiamo concordare sulla espressione di un voto favorevole in ordine al disegno di legge di assestamento per il In conclusione, intendo approfittare di questa sede per sottolineare la necessità di una più complessiva riforma strutturale della procedura di esame dei documenti di bilancio che consenta al Parlamento, per il tramite dei

Grazie, signor Presidente. molto rapidamente devo dire che l'insieme dei documenti che stiamo esaminando smentisce - direi in maniera piuttosto clamorosa - gli assunti del Governo.

è dovuto correre ai ripari, durante la sessione dell'assestamento e del rendiconto alla Camera dei deputati, perché ha dovuto accertare ben 22 miliardi di maggiori commento la facezia del presidente del Consiglio Prodi il quale riferiva che quei miliardi di entrate fossero di pertinenza di questo Governo.

del Governo precedente. Si badi: voci avvertite della maggioranza hanno detto che una delle più probabili cause di quelle maggiori entrate, specie nella parte strutturale che ammonta ad oltre 5 miliardi (tale è ritenuta dal Governo), sia attribuibile ad emersione di materia imponibile grazie alla politica fiscale del precedente Governo. Ciò significa che noi eravamo un'alternativa a questa politica fiscale: oggi il Governo aumenta le tasse; noi non aumentavamo le tasse, anzi abbassavamo le aliquote, ma favorivamo emersione di base imponibile. È qui, nelle cifre e nei dati, la verità sui fatti che hanno interessato in questi anni la manovra finanziaria dei nostri Governi ed è qui, in queste cifre, direi l'errore di fondo della politica fiscale di questo Governo che continua ad aumentare le aliquote, così probabilmente favorendo la sottrazione di materia imponibile. Il Governo ha dovuto registrare questo fatto e, naturalmente, ha dovuto sottacere, sia nelle relazioni sia nel dibattito, questo grande, importante dato; ribadisco: è dovuto, in tutta fretta, ricorrere ad un emendamento alla Camera dei deputati perché il dato nemmeno era stato registrato quando questo provvedimento aveva cominciato il suo *iter* parlamentare. al resto, la critica si appunta sempre sulla dinamica della spesa corrente. Posso dire che l'aver mantenuto una dinamica della spesa corrente nei termini in cui l'abbiamo mantenuta è stato uno sforzo serio in presenza di gravi difficoltà di crescita del Paese, quali quelle che si sono evidenziate a causa di fatti politici noti e di rilievo durante il quinquennio del nostro Governo. Questo è il punto politico di fondo che ci impone una valutazione critica dell'assestamento, così come configurato dal Governo e che i fatti hanno smentito.

sarebbe logico che l'assestamento registrasse anche le minori entrate dovute alla sentenza della Corte di giustizia europea sull'IVA degli autoveicoli.

non espressamente prevista la necessità di assestare una cifra solo per competenza, nella scorsa legislatura, con riferimento ad un provvedimento che stava particolarmente a cuore all'allora maggioranza (quello sulla previdenza agricola),

Per questo ho riproposto l'emendamento 1.Tab.1.1: per ricordare che non si possono usare due strumenti diversi a fronte della stessa situazione.

la minore entrata di 3 miliardi e 700 milioni è relativa al 2006, a regime, e dunque andava registrata nell'assestamento.

una manovra di bilancio di rilevantissima entità: parliamo di 3 miliardi e 700 milioni di euro. La seconda è che, laddove si dovesse adottare un provvedimento amministrativo, il Governo avrebbe dovuto comunicare al

come nella Nota di aggiornamento, sono visibili le verità che questo Governo molte volte ha taciuto o addirittura nascosto agli italiani. Avevamo dato vita ad una politica fiscale che favoriva l'emersione di base imponibile e abbassava le aliquote. L'attuale Governo

comunico che, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, le seguenti Commissioni sono convocate mercoledì 25 ottobre 2006, presso il Palazzo di San Macuto, per procedere alla propria costituzione: Commissione parlamentare per le questioni regionali, alle ore 13,45; Commissione parlamentare per l'infanzia, alle ore 14,30; Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di EUROPOL, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, alle ore 14,30; Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, alle ore 15,15; Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori, di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, alle ore 15,15.